ma come Presidente del Senato, così come alle altre istituzioni, è la seguente: «La stampa ha dato recentemente notizia di dichiarazioni rese da taluni Ministri della Repubblica, e da un Sottosegretario, dalle quali si evince la considerazione in cui costoro tengono

«Nell'indifferente silenzio delle Istituzioni ed in assenza di qualsiasi smentita - che, per essere credibile, sarebbe dovuta immediatamente intervenire con la nettezza ed il risalto consoni alla inaudita gravità delle dichiarazioni - non posso che rassegnare le mie dimissioni da Giudice costituzionale, a tutela, quanto meno, della mia dignità personale». Come sapete e come è stato comunicato da tutti i mezzi di stampa, vi è stato ieri il rigetto unanime

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento nasce da una lunga ed articolata riflessione che si è sviluppata non soltanto ed esclusivamente all'interno delle Aule parlamentari, ma soprattutto del Paese nell'ambito di una serie di eventi, per certi versi anche drammatici, che hanno segnato il calcio italiano in questi ultimi mesi, ma soprattutto alla luce di una serie di riflessioni

In effetti, ormai il calcio in Italia ha un forte valore simbolico, soprattutto un crescente peso di natura economica e al tempo stesso finanziaria.

con una crescita costante in termini di fatturati delle società alla quale però si affianca, in maniera direi pericolosa, un indebitamento progressivo che ha finito per accumularsi durante gli ultimi anni. Alla luce di questi dati, l'importanza del calcio professionistico appare ormai tale che tutto ciò che si sviluppa all'interno di questo settore finisce in qualche maniera per condizionare l'intero sport italiano.

ripetutamente contesi e poi assegnati in maniera diversa rispetto a quanto il campo aveva determinato; gli scandali hanno fatto per certi versi di Calciopoli una piccola nuova Tangentopoli. Come ha reagito la piazza, come ha reagito la tifoseria, quella grande schiera di milioni di tifosi che fanno del calcio il loro punto di riferimento domenicale?

ingannato, in qualche caso defraudato di un punto di riferimento tradizionale: la correttezza della competizione sportiva. È una sensazione che nemmeno la vittoria dei mondiali di calcio, celebrata dal Paese con particolare dovizia di entusiasmo e partecipazione, ha finito per annullare. Cosa sono oggi le società di calcio più importanti? Sono dei veri centri di potere, che hanno dimostrato, in qualche caso e in qualche momento,

presenza corruttiva all'interno di un determinato settore. Se in

per quanto riguarda il concetto di società sportive professionistiche a fini di lucro, la loro quotazione in Borsa, che ha rappresentato un altro limite oggettivo rispetto a società i cui bilanci non sempre erano chiari, e, al tempo stesso, gli equilibri collegati alla vendita di diritti radiotelevisivi, rispetto ai quali non c'è stata vera concorrenza di mercato,

finendo inevitabilmente per condizionare il *budget* annuale e quindi la possibilità di sviluppare una presenza di

ormai semplici *sparring partner* di un processo al quale partecipano in presa diretta e rispetto al quale raccolgono però quasi ed esclusivamente le briciole.

Abbiamo tentato di evitare l'accentuazione del divario tra società sportive con maggiore e minore disponibilità economica, anche perché abbiamo ritenuto che ciò avrebbe finito fatalmente, con il passare del tempo, per annullare ogni valenza competitiva delle manifestazioni sportive,

tutti coloro che hanno avuto modo di partecipare al dibattito, ma soprattutto alla lunga serie di audizioni che ha caratterizzato la fase di analisi.

orientarsi nell'ambito di tutti gli attori del processo collegato all'emittenza radiotelevisiva a livello locale e nazionale, per poi allargarsi a tutti i soggetti che oggi producono informazione di natura televisiva e ovviamente collegata ai *new media*, abbiamo cercato di valutare come

i diritti di cronaca delle grandi *holding* televisive, ma anche, e questo è un dato che è stato recuperato puntualmente (ne approfitto

le TV locali, con particolare riferimento alle serie minori. Nel passato - lo dicevamo ieri nel corso di uno specifico incontro sull'argomento - abbiamo troppo spesso assistito addirittura ad

una sorta di distorsio,ne che finiva inevitabilmente per ricadere sull'emittenza locale, rispetto alla quale questo provvedimento tende finalmente a porre in essere in qualche maniera - direi in maniera precisa, per certi versi - un primo utile intervento. L'ultimo commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, l'amico Luca Pancalli, sottolineava come l'unico importante obiettivo per il calcio italiano fosse quello di riportare serenità all'interno di un ambiente che doveva ritrovare la capacità di dialogo da parte di tutte le sue componenti.

la capacità di seguire i propri campioni, di seguirne i gesti, di ricordarne i *goal*. Credo che un provvedimento come questo riesca soprattutto a ridare ottimismo al pianeta calcio e a tutti gli appassionati, perché finisce inevitabilmente per far ritrovare anche la logica di una competitività che in questi anni probabilmente è mancata.

introducendo inevitabilmente un importante deterrente contro i meccanismi che hanno caratterizzato la

di stabilire un equilibrio di natura competitiva tra tutti i soggetti interessati finisce per sviluppare, attraverso questo provvedimento, un complesso di misure che mi sembra possano utilmente intervenire sulla trasparenza e sull'efficienza del mercato. Il ministro Melandri ha sottolineato più volte come il calcio e lo sport più in generale abbiano acquisito progressivamente in Italia una dimensione di natura sociale ed educativa più vasta rispetto a quella di alcuni anni fa. Noi condividiamo questa impostazione e riteniamo che anche la maggiore diffusione dell'evento sportivo possa costituire un momento educativo più alto, in grado di informare meglio,

realtà che troppo spesso sono state smarrite, direi tradite, all'interno del sistema dello sport italiano. Dicevamo che la distorsione del mercato era evidente ai nostri occhi. Ritenevamo che la titolarità dei diritti non centralizzata, così come si era manifestata nell'ambito degli anni scorsi, fosse oggettivamente un chiaro condizionamento che,

il nuovo meccanismo introdotto all'interno di questo provvedimento, legato ad una commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto che organizza le competizioni sportive stabilendo una regolamentazione corretta ed omogenea del settore, rappresenta un passo in avanti importante e direi decisivo. Del resto, anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - ricordo sotto questo aspetto un'indagine conoscitiva proposta dall'*Antitrust* sul settore legato al calcio professionistico hanno rilevato questa sperequazione sui criteri di vendita dei diritti con penalizzazioni forti e chiare che hanno caratterizzato il sistema calcio in questi ultimi anni. La capacità di gestire in maniera libera, attraverso la vendita centralizzata, sviluppa meccanismi competitivi nuovi e soprattutto recepisce in termini chiari un'esigenza che si era già posta nell'ambito di questi ultimi anni.

Il concetto collegato alle piattaforme in uso, la necessità di garantire la presenza di più operatori che possano impedire le alterazioni di mercato, la capacità di evitare distorsioni di logiche competitive che siano in grado di produrre negative ripercussioni sull'utenza, privandola - come abbiamo detto precedentemente - di una serie di diritti collegati all'informazione: ecco alcuni dei temi più vivi ai quali fa riferimento questo provvedimento.

e riteniamo che gli strumenti che abbiamo individuato siano equilibrati normativamente perché permettono di sviluppare in maniera organica una disciplina, su una materia come quella dei diritti delle trasmissioni televisive, che si muove finalmente su una base di equità, di ragionevolezza, di leale competizione ma soprattutto di trasparenza, Infatti, su questo piano credo che il provvedimento recuperi in maniera oggettiva una realtà di mercato aperta nella quale ogni soggetto può ritrovare le ragioni della sua presenza, ma soprattutto può recuperare, a livello delle emittenti locali e più lontane, il concetto di un'*audience* legata fatalmente alla propria società, alla propria squadra, alla propria tifoseria. Con questo spirito abbiamo lavorato, su queste basi abbiamo costruito il nostro impegno, cercando di disegnare un percorso per certi versi faticoso ma certamente di straordinaria attualità, disponibili come siamo, naturalmente, a valutare ancora tutti gli ulteriori correttivi che il Parlamento,

ma le due Commissioni del Senato - voglio sottolinearlo - hanno svolto un approfondimento ulteriore che ci ha permesso precisazioni importanti e modifiche utili e significative. Dico ciò volentieri oltre che come relatore

il senatore Scalera, dalle audizioni svolte nonché dagli interventi delle diverse componenti parlamentari - anche questo mi sembra un punto significativo

Dal nostro confronto viene confermata la volontà e la proposta di una riforma profonda dell'ordinamento della disciplina dei diritti televisivi negli eventi sportivi e questo secondo due assi fondamentali. In primo luogo, si superano la vendita e la contrattazione da parte dei singoli *club* e si introduce la vendita centralizzata e collettiva;

una mutualità accentuata, un'attenzione ai vivai, altro punto fondamentale che abbiamo posto e su cui ci siamo soffermati e sul quale abbiamo ottenuto un larghissimo consenso da tutte le associazioni e gli enti sportivi auditi

Il secondo asse è la grandissima attenzione prestata e le misure chiare presenti nel provvedimento contro la formazione di situazioni monopolistiche tra gli operatori delle comunicazioni.

una situazione come quella attuale di grave squilibrio competitivo nei campionati anche a causa della redistribuzione delle risorse. Poche squadre prendono il massimo della torta dei diritti televisivi mentre le altre, pur giocando negli stessi campionati, o meglio nello stesso campionato,

non può più essere tollerata l'affermazione di posizioni monopolistiche che tra l'altro penalizzano le nuove tecnologie, le piattaforme emergenti, l'informazione locale, il diritto di informazione. Anche questi sono punti che ci sono stati sottolineati come temi su cui sviluppare una grande attenzione di riforma. Vorrei sottolineare che a mio avviso non ci troviamo a questo punto negativo solamente per il cambiamento della normativa effettuato nel 1999,

se questo provvedimento riuscirà, o se mai riusciremo - come del resto è necessario - far registrare elementi di trasparenza e di legalità e a far saltare i meccanismi di corruzione che probabilmente esistono ancora, anche dopo Calciopoli, nel mondo del calcio e in altri sport. Non so se si riuscirà a far saltare questo meccanismo deteriore; certo è che il Governo, con il provvedimento contro la violenza

da parte dell'Osservatorio del Ministero dell'interno. Ho letto che è questione di dettaglio, ma guardate che queste cose possono portare a esasperazione, piuttosto che a a salvaguardare un clima sereno sugli spalti degli stadi. Mi piacerebbe che su questo aspetto si corrispondesse davvero alla lettera alla legge che è stata approvata. Ritorno al punto dicendo che in Commissione, come il senatore Scalera sottolineava, abbiamo, mi pare, contribuito a precisare, a migliorare e a definire un cambiamento significativo nel provvedimento che ci veniva proposto, per quanto si possa e si debba fare in una legge delega; anche questa della

poi le questioni più specifiche, di dettaglio, siano pienamente aggiornate al momento della loro applicazione.

governo di questa partita così delicata e importante. Altrettanto significativo è l'aver sottolineato la necessità di sostegni di sostegni alle piattaforme emergenti, al fine di far crescere la presenza plurale degli strumenti informativi e della comunicazione in questo campo come in altri.

non dico rapidissimo, ma in tempi equi. Mi sembra molto importante l'aver definito come, nel quadro di una responsabilizzazione delle società

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la delega sui diritti TV di cui oggi discutiamo consente di affrontare con decisione una situazione che si era fatta ormai insostenibile: la vendita individuale dei diritti TV nello sport e in particolare nel calcio in questi anni ha fatto male allo spirito sportivo di quello che è un fenomeno sociale di estrema importanza. Affrontiamo questo passaggio con la consapevolezza che la presenza pervasiva, nei palinsesti televisivi, del calcio ha modificato la natura di questo sport, portando elementi positivi, come la più ampia diffusione di quello che è un vero e proprio evento collettivo, ma introducendo anche elementi estremamente negativi, come la frammentazione del calendario e la crescita senza limite delle spese per le società sportive. Con questo primo intervento noi riaffermiamo il principio di mutualità tra le diverse squadre, elemento fondamentale per una sana e corretta competizione, ma soprattutto riaffermiamo come l'attività sportiva, anche professionistica, prima ancora che un'attività di rilevanza economica sia un fenomeno identitario e culturale. La delega che affrontiamo in questa sede ci pone una discussione di ordine generale che spesso ha fatto e fa visita nelle riflessioni dei soggetti più diversi: lo sport, e specificamente il calcio, è prioritariamente un'attività sportiva o un'attività economica? Questo interrogativo è apparso come evidente quando il presidente della Lega Calcio, alcune settimane fa, di fronte alla paventata chiusura degli stadi per più di una giornata, ha detto con chiarezza che lo spettacolo sarebbe dovuto continuare e ha utilizzato un parallelismo molto ardito tra l'attività calcistica e una grande azienda. Di fronte alla morte dell'ispettore Raciti e alle vicende che a quell'evento drammatico sono seguite, questa questione si è posta con evidenza, ma è la stessa questione che ha fatto da sottofondo ai lavori delle Commissioni. L'attività sportiva, fosse anche a livello professionistico, è solo un mercato e un'industria come tante altre? Credo che questa ipotesi, praticata prima ancora che dichiarata negli ultimi anni, abbia prodotto effetti gravi e profondi nella società. Tutti noi abbiamo sempre ritenuto che lo sport avesse una grande valenza educativa e identitaria: innanzi tutto educativa, al punto che le lezioni di educazione fisica sono, nelle scuole di tutti gli ordini e gradi, affrontate con pari dignità rispetto alle altre materie. Ma lo sport, è evidente, ha anche un grande peso nella definizione identitaria dei popoli: si pensi solo all'orgoglio nella recente vittoria al campionato mondiale di calcio e ai tantissimi esempi che si potrebbero fare al riguardo. Invece, nella pratica reale di quest'ultima fase, si è voluto fare dello sport unicamente un mercato. Faccio solo alcuni esempi. Il primo evidente è l'aumento del numero degli eventi sportivi, in nome della vendibilità di prodotti televisivi; siamo ormai a campionati spezzatino nei quali logiche diverse da quella del profitto, fosse anche la sicurezza negli stadi, non sono ammesse. Un secondo esempio è la crescita esponenziale di sostanze dopanti. Il *doping* non è soltanto un additivo chimico per la conquista della vittoria, ma anche l'unico modo di rendere in serie le prestazioni che, di fronte ad investimenti ed aspettative di profitto, non possono essere delegate all'estro dell'atleta. Il terzo, che è sotto gli occhi di tutti, è il rapporto malato tra tifo organizzato, anche violento, e società, un rapporto visibilmente macchiato da interessi prioritariamente economici, dai biglietti omaggio al *merchandising*. Il quarto esempio è quello degli eccessi nella compravendita di giocatori e sportivi in genere, i cui costi sono lievitati negli ultimi anni. Il punto che solleviamo non è una certa nostalgia per i bei tempi andati, ma la consapevolezza che uno sport inteso unicamente come mercato, in causa degli enormi effetti sociali di questo fenomeno, è un danno per il tessuto sociale del Paese. E non possiamo che sottolineare con soddisfazione il richiamo, presente nel provvedimento che stiamo esaminando, alla dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza, che definisce lo sport «un'attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali», nonché «un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole». Se questo è il contesto nel quale agiamo, credo che questo primo atto normativo debba essere rivendicato come un elemento di moralizzazione della sport. Ritornare alla contrattazione collettiva dei diritti e fare di questa procedura la via maestra per tutto lo sport e per tutte le piattaforme è un primo gesto di affermazione che lo sport non è un mercato. Se l'effetto di questa norma sarà che alcune squadre non potranno più acquistare campioni da 50 milioni di euro, non ci sembra questo un grande danno; anzi forse sarebbero maturi i tempi per avviare una profonda riflessione su formule di *price cap* in grado di calmierare gli stipendi dei giocatori. Per questo reputo incomprensibili le obiezioni di chi sostiene che la logica mutualistica sia inadatta a questo comparto: il punto è proprio che le logiche del mercato forse sono in grado di garantire profitti ad alcuni, ma snaturano il senso profondo del fenomeno sportivo. Proprio a partire da queste premesse salutiamo con soddisfazione il lavoro svolto in Commissione, che ha reso la proposta del Governo più puntuale e incisiva nella regolazione di questo mercato e nella funzione che questo tipo di contenuto può avere nello sviluppo di un sistema di maggior competizione tra gli attori e le piattaforme che operano nella trasmissione dei contenuti. Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione tecnologica, della quale ancora non è noto l'esito: dalle televisioni via cavo che trovano in Internet un alleato naturale, con la cosiddetta IPTV, fino al satellite e al digitale terrestre sono svariate le piattaforme che si candidano a soppiantare la tradizionale televisione per come l'abbiamo conosciuta fino ad ora. E proprio il calcio è spesso l'elemento trainante di questa competizione tecnologica. Questo provvedimento, migliorato in Commissione, consente una competizione tra pari, in un contesto in cui il duopolio televisivo rischia di far arenare qualunque significativa innovazione. A fianco a questo, l'altro aspetto rilevante è quello della destinazione delle risorse allo sviluppo dei vivai e alla sicurezza delle strutture sportive. Dopo il dibattito su chi dovesse farsi carico delle ristrutturazioni degli stadi, vividamente rappresentato dal decreto contro la violenza degli stadi, oggi siamo in grado di indicare una risposta chiara. La domanda «Chi paga?» per la sicurezza negli stadi e per gli interventi strutturali è stata copiosamente ripetuta: abbiamo assistito addirittura a tabelle sui quotidiani di quanto sarebbe costato ogni intervento; ed è un problema reale, che non può essere risolto con un'alzata di spalle. Se si assume il principio che le risorse dei diritti TV sono risorse innanzitutto del calcio e non solo delle singole società, come si evince chiaramente dalla contitolarità dei diritti di sfruttamento, destinare parte di queste risorse al bene comune del movimento calcistico e quindi alla sicurezza negli stadi sarebbe un intervento utile e positivo. In questo senso, un intervento unitario rivolto a tutto lo sport non agevola, visto che ad esempio parlare di sicurezza nel mondo del *rugby* o del calcio o addirittura negli sport motoristici è cosa assolutamente differente. Ma proprio la flessibilità dello strumento della delega, con l'emendamento che è stato accolto in Commissione, consentirà al Governo di operare con puntualità. Mutualità, trasparenza e moralità nella gestione delle principali entrate del mondo sportivo sono stati i princìpi cardine che abbiamo assunto nel proficuo lavoro della Commissione: sono questi gli unici princìpi che consentono di riconoscere davvero quel carattere educativo e di passione che milioni di cittadini affidano allo sport.